solo poco più di 200 corrotti e corruttori sono nelle carceri italiane. Questo mostra la grande importanza di proseguire la lotta alla corruzione. Il mio voto sarà favorevole, anche se avrei preferito un testo più integralmente in linea con la formulazione del presidente Grasso. Vorrei aggiungere che mai, nella lotta alla corruzione, un provvedimento può dirsi definitivo. Tra le strategie che ancora credo debbano essere valorizzate in Italia per favorire una maggiore efficacia nella lotta alla corruzione c'è anche quella, che può sembrare estranea alla cultura italiana, di dare un ruolo importante ai denunzianti civici, come vengono a volte denominati, o ai *whistleblower*. La corruzione è in fondo un fenomeno di collusione e la denuncia, che una certa tradizione culturale italiana è portata a vedere come delazione, può fornire un contributo estremamente importante alla lotta contro la corruzione. In tutto il mondo, ormai, per un altro comportamento collusivo, quello dei cartelli in violazione degli interessi dei consumatori, si fa ricorso in modo sistematico all'utilizzo di queste denunce, assicurando benefici giuridici a chi fondatamente le formula. formulare una raccomandazione che contiene anche un rilievo critico al Governo, e in particolare al Presidente del Consiglio. Nel governare, un Governo non solo indirizza il Paese e conduce le politiche, ma anche - che lo voglia o no - trasmette valori, educa i cittadini, dà esempi. Un aspetto che apprezzo del presidente Renzi è proprio il fatto di sottolineare spesso che per conseguire determinati obiettivi, dalla crescita economica alla coesione sociale, occorra anche un cambiamento di alcuni tratti della mentalità di noi cittadini italiani. Ne sono sempre stato convinto anch'io. Occorre in particolare instillare un maggior rispetto per la legalità e una maggiore sanzione sociale o stigma nei confronti di chi viola la legge a danno della collettività.

sotto questo profilo, io sono stato in passato critico nei confronti di un accordo politico stipulato all'inizio di questa legislatura e vorrei, con grande serenità,

Del resto, ho più volte detto pubblicamente che, pur essendo i provvedimenti di clemenza di competenza esclusiva del Capo dello Stato, non avrei trovato fuori luogo se questi fossero stati o fossero presi in considerazione con riferimento al presidente Berlusconi. Però, in termini impersonali, prescindendo dalla persona, si è verificato che il Presidente del Consiglio ha stipulato un patto politico fondamentale con una persona condannata in terzo grado per un reato fiscale e non più parte del Parlamento per una conseguenza legale di tale condanna. Tutto potrà cambiare, ma rimane il fatto che il Presidente del Consiglio ha dato al Paese l'impressione di considerare più importante avere un appoggio per determinate riforme costituzionali o per una modifica della legge elettorale che non trasmettere un forte significato di lotta contro l'evasione e contro la corruzione. Ecco, credo che in queste Aule noi spesso ci convinciamo che le riforme costituzionali e le riforme istituzionali

questo farebbe veramente fiorire l'Italia. Quindi approvo con convinzione questo provvedimento e mi auguro che mai più vengano dati segnali che, sul piano dell'educazione di fatto dei cittadini, possano dare l'impressione di non mettere in primissimo piano l'interesse della lotta all'evasione e della lotta alla corruzione.

C'è stato un ampio dibattito, che ha evidenziato sicuramente delle criticità. Non da ultimo, c'è stato un percorso abbastanza articolato di questo disegno di legge, ha visto l'assegnazione alla Commissione giustizia da moltissimo tempo; esso poi è stato lungamente trattato ed ha affrontato sicuramente delle curve un po' strette. Andiamo a parlare di un tema che purtroppo diventa di interesse in Italia, visto che nel nostro Paese la corruzione rappresenta ancora oggi un indice di particolare difficoltà.

fa pensare quasi con una forma di nostalgia al vecchio sistema obsoleto delle mazzette, un ingenuo corpo del reato, quando oggi si assiste invece a fenomeni di corruzione ben più complessi, ben più complessi, in cui il sistema stesso e la stessa organizzazione di tipo normativo arrivano quasi a dare le chiavi della cassaforte direttamente al ladro.

comporta delle conseguenze sulla stessa alterazione della concorrenza. Infatti, per certi versi, chi è capace di corrompere può avere anche vie più strategiche rispetto ad altri. Dobbiamo anche pensare a tutta una serie di costi che vengono ad incidere, e che sono una conseguenza del fenomeno della corruzione. Ci sono costi diretti, che sono stati evidenziati anche dalla stessa Corte dei conti, ma, soprattutto, costi economici indiretti: costi che vengono ad incrementare, per certi versi, anche gli importi delle opere pubbliche, derivanti dai ritardi stessi della definizione di alcune pratiche amministrative. Dobbiamo pensare tutti a quali sono i costi veri che vengono ad incidere su tutto il sistema Italia. Costi conseguenti al disvalore totale che viene prodotto nei confronti della stessa pubblica amministrazione,

bene, ad esempio, l'introduzione dell'ipotesi della riparazione pecuniaria, imponendo, quindi, che vi sia un ristoro rispetto a quanto viene commesso, una restituzione del maltolto. Bene anche l'ipotesi del falso in bilancio nella sua genericità, in quanto viene ad aggravare la previsione normativa attualmente contenuta nel codice. Ma quello che ci domandiamo è se questo provvedimento possa essere

come una sorta di panacea per il male della corruzione, e questo è un grave errore che sta commettendo sicuramente il vostro presidente Renzi quando viene a parlare, amplificando gli effetti di queste previsioni normative. In realtà, non è una panacea per la corruzione. La corruzione non nasce solo da una previsione; non può essere mortificata e combattuta solo con aumenti di pene, perché la corruzione deriva anche da un modo di operare. Vi sono mali nell'Italia che saranno difficilmente superabili, a questo punto. Vi è un problema nella burocrazia; un problema che riguarda la lunghezza dei procedimenti amministrativi e la laboriosità degli stessi;

Sotto questo profilo nulla è stato fatto. Nulla è stato previsto in questo provvedimento. Nulla è stato previsto anche per quanto riguarda settori estremamente delicati, che, purtroppo, sono balzati anche ai disonori delle cronache.

Vi sono problemi che riguardano la trasparenza stessa dell'attività amministrativa. Quindi, noi ci diciamo che forse, visto che c'è stato il tempo di meditazione su questo provvedimento, si poteva approfittare dell'occasione

del Governo e della maggioranza. Nel provvedimento al nostro esame sono stati previsti degli aumenti di pena che alcuni colleghi hanno evidenziato come probabilmente anche poco inquadrati dal punto di vista sistematico nella normativa stessa. tuttavia, che parlate in questo momento di aumenti di pena, come a voler essere voi i paladini, perché dobbiamo ricordare che nel frattempo, negli ultimi due anni, c'è stata una sequenza di provvedimenti che hanno previsto

tutti dei paladini della grande giustizia, quando poi alla fine ci troviamo con un sistema normativo e della giustizia come il nostro, un sistema di benefici a favore dei criminali. Come facciamo poi a vedere effettivamente applicate queste

credenze popolari su donne guaritrici, che magari con il piatto cercano di guarire una certa malattia: è il percepito che poi porta ovviamente ad estreme conseguenze, alla morte del paziente. Lei sa anche perfettamente che in una malattia "banale" come il diabete, che si cura con l'insulina, una dose eccessiva, una dose da cavallo porta a morte il paziente. Le ho fatto questi due esempi perché l'evidenza scientifica parte da dati concreti

profilo sociale, morale e finanziario è una realtà inconfutabile. Condurre una battaglia dura contro fenomeni odiosi, che imperversano

metaforici, a mo' di parabola, per far capire che non si può giocare con le cose serie e lavorare di fantasia, bisogna tornare alla realtà, la prevenzione è sempre migliore della cura

ed ebrei. Dunque, in scia con un populismo che non va oltre il proprio naso, si è ritenuto di procedere con un inasprimento delle pene, sia minime

con fermezza e celerità a fenomeni così odiosi, mi domando che senso abbia darsi una *dead-line* a vent'anni, quando ci sarebbe invece bisogno di intervenire subito, senza ulteriori indugi: come ho avuto modo di dire attraverso un emendamento, facciamo dei tribunali speciali o specifici, come si fa in chirurgia, in cui un ortopedico non cura problemi ginecologici e viceversa. Aumentare le pene non è, a mio avviso, un deterrente valido. Il problema c'è, è serio e pertanto va estirpato. Servono misure che impattano in maniera forte e decisa contro la corruzione, ma da subito perché siamo già in ritardo. Gli *spot* non servono e, ahimè, in questo testo ve ne sono fin troppi, tanto da costituire Mettiamo in galera i corrotti, si grida da più parti: giusto! Dopo averli messi in carcere, buttiamo la chiave: va bene! Diamo la possibilità di punire Ma dov'è la parte in cui in cui si combattono tali delitti? Non credo che gli italiani siano animati da uno spirito di vendetta a tutti i costi e comunque la nostra Costituzione non lo prevede. Credo che essi chiedano il superamento di certi fenomeni contrari alla legge, alla loro stessa tutela. tutela. Credo vogliano vedere garantiti i propri diritti e che sarebbero più contenti di sapere che le leggi vengono rispettate e non che i colpevoli, che vanno puniti senza se e senza ma, vivano lunghi e dolorosi travagli. Alla luce di quanto sempre più frequentemente emerge in tema di crimini contro la pubblica amministrazione, credo non si possa più prescindere da interventi a priori, senza agire solo con come quelli al vaglio di questa Assemblea. Occorre debellare questo malcostume prevenendolo, se si vuole riuscire a voltare veramente pagina. L'abbiamo già fatto con la legge Severino, nel 2012, e non è servito a nulla; lo rifacciamo oggi e non servirà a nulla. È necessario

prevenzione, quindi, come cometa da seguire al fine di limitare quanto più possibile l'eventualità stessa del verificarsi di scandali, qualora si accerti siano effettivamente tali, come quelli che sempre più spesso assurgono agli onori della cronaca. ancora un volta, la linea guida sembra essere la mera repressione nuda e cruda; repressione che certamente ci deve essere - e ci mancherebbe altro! - ma che non può essere utilizzata come un dissuasore. Credo ancora nel legiferare in maniera da limitare la possibilità stessa di Lo Stato ha infatti il compito di reprimere comportamenti contrari al proprio impianto normativo, ma anche quello di prevenirli. Le leggi servono non soltanto a punire chi le infrange, ma anche a limitare in partenza comportamenti contrari

in cui la morale dei potenti di turno la fa da padrona. Ed allora, si pone nel mirino questo piuttosto che quel fenomeno e si tira dritti, mossi dalla convinzione che quello sia il male assoluto, da combattere con tutti i mezzi. Infine, signor Presidente,

Signor Presidente, colleghi, signori del Governo,

non rinunciando però ad esprimere qualche valutazione rispetto alle problematiche che abbiamo affrontato, verso le quali pensiamo si debba agire anche con altri strumenti e non soltanto con la repressione penale. in primo luogo, all'avvio e all'attuazione di controlli preventivi efficaci e mirati rispetto ai luoghi ed alle aree dove l'attività illegale si manifesta con maggiori dimensione e preoccupazione. Il controllo preventivo consente di intervenire prima che il danno sia arrecato e che sia stato portato all'estremo compimento, nei confronti della pubblica amministrazione e, più in generale, della cittadinanza tutta, che attraverso il fenomeno corruttivo vede limitare la capacità del Governo di realizzare opere, di cambiare profondamente e modernizzare il nostro Paese. controlli preventivi avendo anche il coraggio di andare a rivedere l'esperienza del passato, non tutta da cancellare: mi riferisco, in particolare, alle attività che i segretari comunali hanno svolto nel passato; i comitati regionali di controllo, seppure con i loro limiti, esercitavano comunque un'azione preventiva che, essendo venuto meno, ha provocato una deriva, una slavina di comportamenti illegali. Purtroppo il controllo oggi è affidato soltanto alla magistratura penale e sappiamo che quando la magistratura penale si muove vuol dire che il danno, purtroppo, è stato arrecato. Vorrei richiamare l'attenzione anche su una serie di questioni che abbiamo posto come Gruppo e che non hanno trovato risposta positiva da parte del Governo e del relatore. mi fa piacere che il senatore Monti ne abbia parlato, sottolineo il ruolo di una collaborazione civica che nelle pubbliche amministrazioni si deve anche estrinsecare attraverso la denuncia che il pubblico funzionario, di fronte a comportamenti illeciti, nella sua responsabilità civica e non soltanto di pubblico ufficiale, compie segnalando all'autorità competente il fatto. Da questo punto di vista, credo che sarebbe stato utile prevedere forme di riservatezza e di tutela onde non non metterlo in una condizione di disagio all'interno del proprio ambiente di lavoro. È necessario quindi sviluppare con maggiore attenzione una garanzia nei confronti delle indagini. Ho presentato un emendamento che si legava alla riservatezza dell'informatore e tendeva a sanzionare con maggiore il comportamento di elementi che concorrono all'attività giudiziaria nelle varie fasi e diventano uno strumento di comunicazione verso l'esterno, anche con la finalità di creare un giudizio negativo nei confronti di cittadini che, invece, non hanno nessuna responsabilità giudiziaria e che, pertanto, dovrebbero rimanere estranei all'azione della magistratura. È un limite, a mio avviso, il fatto di avere accettato la corruzione in atti giudiziari, ma non avere accettato in maniera altrettanto necessaria la concussione in atti giudiziari. Fa un po' specie il fatto che, di queste due fattispecie di reato, uno abbia un riconoscimento anche nel comportamento illecito del magistrato e l'altra no, come se l'atteggiamento concussorio di un operatore della giustizia non possa accadere: una sorta di presunzione di infallibilità rispetto a un comportamento che, invece, e purtroppo, come rileviamo dalle cronache, si registra. di questioni che ci fanno esprimere un giudizio positivo ma non entusiastico di questo provvedimento, perché l'aumento delle pene non è garanzia di efficacia dell'azione di contrasto. Noi abbiamo bisogno di certezza delle pene, di rapidità delle sentenze e dei processi, affinché diano la consapevolezza immediata che chi commette un comportamento illecito possa arrivare rapidamente a una verifica della sua liceità o meno, e in modo che se c'è stato un comportamento illegale arrivi subito la sentenza di condanna.

non soltanto per quanto riguarda le società quotate, sarebbe stata forse utile una differenziazione tra le piccole imprese e quelle medio-grandi. Non c'è soltanto una questione di principio (credo che debba valere per tutti, grandi e piccoli), ma c'è una questione di quantità che diventa elemento sostanziale, perché il danno arrecato da un piccolo imprenditore alla comunità è molto limitato, almeno

alla trasparenza e alla concorrenza della nostra economia. Quindi un diverso scadenzamento di questa problematica sarebbe stata più utile. In ultimo, signor Presidente, signor Ministro, probabilmente sarebbe in sede di valutazione del falso in bilancio e degli atti connessi, criteri espliciti di valutazione, onde non lasciare non tanto al magistrato al perito che stila l'elemento tecnico l'arbitrarietà che noi sappiamo esserci all'interno di queste problematiche di bilancio. Francamente, ciò avrebbe dato maggior certezza di comportamenti ai cittadini e anche all'autorità chiamata a decidere. Concludendo, signor Presidente, signor Ministro, io credo che noi oggi stiamo realizzando un passo in avanti. Io sono un riformista e sono convinto che vale la pena percorrere un passo dopo l'altro, avendo però sullo sfondo un principio di carattere generale che è stato messo a dura prova dal nostro ordinamento; aumentare le pene, aumentare la prescrizione derivante, aumentare la prescrizione *sic et simpliciter* non è una buona risposta alle problematiche giudiziarie del nostro Paese. Dovremmo potenziare gli apparati, arrivare rapidamente alle sentenze, arrivare a sentenze certe e non biunivoche a seconda del perito o del collegio giudicante, pur restando fermo il principio costituzionale della libera discrezione del magistrato in funzione della valutazione dei fatti e delle norme collegate.

finalmente arriviamo alla fine di un percorso che è stato estremamente travagliato; un percorso riguardante una materia che forse avrebbe meritato una riflessione più omogenea e unitaria. Forse quel disegno di legge che noi avevamo avevamo in discussione in Commissione giustizia dall'inizio di questa legislatura avrebbe meritato di dar luogo a una discussione ampia, come quella che c'è stata, ma anche onnicomprensiva;

sia presente nei termini in cui era prevista dal disegno di legge che avevamo qui in discussione. È rimasto l'innalzamento delle pene, che è diventato anzi il nucleo centrale di tutta la parte riguardante i reati contro la pubblica amministrazione;

chi si è messo in questi reati di corruzione, una sorta di dimostrazione della sua buona volontà.

costituzionalità e di giustizia, atteso che se deve passare il principio che abbia una natura rieducativa, forse tale principio deve passare nei confronti di tutti.

di mese in mese, gravata di responsabilità. Tuttavia, alle volte ciò può anche essere pericoloso, perché può spostare su un unico snodo quella che invece deve essere una responsabilità condivisa.

si dice ‑ a una traduzione dall'inglese, che sicuramente sposta il problema da un discorso più ampio (quello che comprende anche le valutazioni)

ha ammesso che qui stiamo producendo una norma che necessiterà di interpretazione ben più di quanto, secondo noi, oggi si dovrebbe fare soprattutto in questa materia. È chiaro che un avvocato cassazionista possa avere una sorta di riflesso pavloviano di fronte alla scelta tra una norma che sia più chiara e un'altra che, invece, apra al tripudio della discussione in Cassazione (che, però, spesso è quella

o alla responsabilità dei giudici quella che secondo noi avrebbe dovuto essere una certezza e una chiarezza, anche per via dell'importanza della fattispecie del falso in bilancio. Chi vuole - e non perdo tempo a richiamarlo - può anche andare a vedere sui giornali

e stime. Questo aspetto è rilevante ma non ci impedirà, in ogni caso, di esprimere un voto positivo sulla globalità di questo disegno di legge, pur essendoci noi astenuti su tutti gli articoli che riguardano il falso in bilancio; non ci impedirà di

dal senatore Monti in apertura.

ad un arricchimento immediato e al potere. Questa responsabilità è del singolo, a tutti i livelli, perché la corruzione può essere di lieve entità solo perché la possibilità di corrompere e di essere corrotti è di lieve entità o la possibilità di falsificare è di lieve entità; ma, in realtà, se fosse nella condizione di poter corrompere per maggiori entità, forse chi l'ha fatto per piccole entità sarebbe disponibile. È una disponibilità che si crea pian piano, nella mancanza del senso della vergogna, nella mancanza della vergogna di presentarsi, poi, di fronte agli altri

invece una cronaca di personaggi pubblici che hanno gravemente mancato. La gravità del loro comportamento è tanto più forte in quanto sono diventati un consolidato esempio di come sia, tutto tutto sommato, non così frequentemente sanzionabile, non così socialmente sanzionabile il loro comportamento. Questa è la cosa che mi fa più effetto. In una cultura della vergogna si attivano dei meccanismi di esclusione sociale che sono quelli che dovrebbe indurre anche a lottare contro la criminalità organizzata e non solo contro i fenomeni corruttivi. È quella sanzione sociale che dovrebbe indurre tutti a desiderare di non frequentare coloro che si sono macchiati di corruzione, quantomeno di non frequentarli pubblicamente, di non dare loro un credito pubblico. A questo aggiungo che

un pezzetto di strada e, forse, comunque quello non più decisivo in un percorso molto più ampio che deve essere quello di una consapevolezza in tutte le procedure amministrative

seppur lo ritiene una tappa di altri interventi dei quali parlerò alla conclusione di questo mio intervento. È un disegno di legge che si muove nella logica del rafforzamento dell'aspetto sanzionatorio e delle pene accessorie. Si guarda ad un inasprimento delle pene e, forse, un po' meno agli atteggiamenti di prevenzione della corruzione, che meriterebbero anche un'analisi più approfondita e che mi auguro il Governo metta in cantiere. Parliamo di un appesantimento dell'efficacia delle pene accessorie, del divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio. Questa sospensione non può essere superiore a cinque anni, mentre prima era di tre.

significativo. Priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, la stessa professione. Sono pene che incidono sulla libertà dell'esercizio professionale ma che in questo caso, sì, esprimono la sanzione e la deterrenza nei confronti del pubblico professionista.

Per il reato di peculato prevediamo l'aumento notevole della pena edittale e, nel caso di corruzione per un atto contrario ai doveri di uffici, anziché innalzare la sola pena edittale più alta siamo intervenuti su quella più bassa: a otto anni passiamo da sei a dieci anni, tanto da essere stati poi costretti, essendo intervenuti troppo o in maniera molto convinta sull'aumento del minimo della pena edittale, a prevedere l'innalzamento dei benefici di legge, pari a due terzi della pena nel caso in cui si voglia collaborare. Ci si è resi conto che l'abbuono solo di un terzo della pena era insufficiente per poter indurre il soggetto ad aspirare ad eventuali benefici di legge che gli potessero consentire la sospensione della pena. Nella concussione abbiamo previsto l'equiparazione importantissima tra il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio perché in effetti non ha senso punire soltanto il primo, il pubblico ufficiale, quando lo stesso comportamento può essere posto in essere anche da un concessionario di pubblico servizio.

con la sentenza di condanna per alcune tipologie di reato contro la pubblica amministrazione viene ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Questa è una svolta epocale nella riforma dei reati contro la pubblica amministrazione. Altra riforma importante il patteggiamento della pena soltanto nel caso di restituzione del corpo del reato, vale a dire dell'oggetto della corruzione. Nello stesso tempo la sospensione condizionale della pena viene subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato. Quindi, non solo patteggiamento ma anche sospensione condizionale della pena.

E lo stesso giudice amministrativo, allorquando si trova a decidere su contenziosi che attengono a lavori pubblici o a pubblici appalti, è tenuto a trasmettere alla commissione per la trasparenza dei pubblici appalti le anomalie che intravede nelle procedure. La riforma, quindi, comincia a coniugare una sinergia di collaborazione tra organismi che collegialmente possono interferire e innervarsi nell'esigenza di una maggiore trasparenza nell'ambito del lavoro della pubblica amministrazione, dell'erogazione dei pubblici servizi e della fruizione di pubblico denaro come compenso per le attività

seppur abbiamo ribadito l'esigenza di intervenire anche sulle procedure finalizzate a prevenire la corruzione. Mi riferisco alla provvista della corruzione, alla costituzione di fondi neri, a maggiori controlli neri, a maggiori controlli sulle gare, sulle fatturazioni, sulle dinamiche di spesa dei soggetti committenti e di quelli appaltatori. Al tempo stesso riteniamo che questo passaggio non possa che essere il primo di una grande riforma della giustizia che attendiamo qui, al Senato, relativamente ai temi della prescrizione e delle intercettazioni. Signor Ministro, lei si è impegnato, allorquando è stato votato il testo sulla prescrizione con la nostra astensione, a modulare nuove proposte su questo aspetto.

non soltanto dei processi ma anche delle indagini, quelle indagini che talvolta sono troppo lunghe e determinano il 60 per cento dei casi di prescrizione dei processi. Ci attendiamo questo anche perché vogliamo vedere con attenzione quale sarà il prodotto finale di questa riforma. Infatti, non siamo convinti che il tema dell'eccessiva anomalia delle prescrizioni prescrizioni si risolva soltanto con la dilatazione dei tempi di prescrizione. Non è questa, secondo noi, la misura esclusiva, non è la sola misura giusta. Ci innamoreremmo di più di sentir parlare di prescrizione delle fasi processuali, in maniera tale da poter incardinare i tempi della giustizia in argomenti e temi che si chiudano in determinati periodi di tempo. Troppo lunghe le indagini, troppo lunghi i processi, troppo lunga la prescrizione. Dobbiamo impedire che il cittadino sia in balia di indagini o processi che durano vent'anni per due ordini di motivi: per evitare che dopo vent'anni la giustizia chieda scusa al cittadino per essersi sbagliata e quindi per evitare che si possa sottoporre a sanzione penale e a una pena una persona che dopo vent'anni è notevolmente cambiata ed è diversa dall'epoca in cui commise il reato. È un'altra persona, che magari si è inserita nella società, ha una famiglia, dei figli e delle aspettative e ha dato quello che doveva dare alla società. società. Altro tema, signor Ministro: ci aspettiamo da lei - e ce lo aspettiamo tutti - uno scatto sul tema delle intercettazioni. È giunto il momento di occuparci di questo argomento, senza nessuna volontà di mettere il bavaglio all'informazione e alla stampa. Io credo che i fatti di questi giorni, i fatti dei precedenti mesi e i fatti dei precedenti anni inducano la classe politica a mettere ordine non tanto all'utilizzo delle intercettazioni come mezzo per accertare la verità, quanto come mezzo di tutela della *privacy* di tanta gente perbene, che si trova schiaffata in prima pagina senza essere indagata, senza rilevanza penale, con un prezzo altissimo che paga in termini di credibilità e dignità Ne va della nostra civiltà, della civiltà del nostro diritto e della civiltà del nostro Paese.

Vorrei semplicemente precisare che, se questa è un'intimidazione che viene fatta nei confronti del Gruppo, non ci riuscirà mai nessuno a fare una cosa del genere. Lo dico con grande pacatezza. Mi permetto di dirlo Faccia parlare il suo Capogruppo, Detto questo, ricordando che, se si trattasse - ma credo che non succederà mai - di andare in galera per difendere gli interessi dei cittadini, saremmo sempre pronti perché non ci

«La corruzione è una nemica della Repubblica. I corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà. Dare loro solidarietà per ragioni di amicizia o di partito significa diventare complici di questi corrotti. Bisogna essere degni del popolo italiano. Non è degno di questo popolo colui che compie atti di disonestà e deve essere colpito senza alcuna considerazione. Guai se qualcuno, per amicizia o solidarietà di partito, dovesse sostenere questi corrotti e difenderli. In questo caso, l'amicizia di partito diventa complicità ed omertà. Deve essere dato il bando a questi disonesti e a questi corrotti, che offendono il popolo italiano, offendono i milioni e milioni di italiani che, pur di vivere onestamente, impongono gravi sacrifici a se stessi e alle loro famiglie. Quindi la legge sia implacabile e inflessibile contro i protagonisti di questi scandali, che danno un esempio veramente degradante al popolo italiano». Queste sono le parole di Sandro Pertini, un Presidente di questa Repubblica degno di questo nome. quello che rileviamo in questo provvedimento è che si tratta di un'ennesima occasione persa, attesa da due anni; un'occasione forse consapevolmente persa persa perché c'è l'assenza di misure concrete e profonde per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione. Non siamo giustizialisti, come a volte qualcuno ci vorrebbe dipingere. Per questo proponevamo non solo misure per punire i corrotti, ma anche misure per prevenire il fenomeno, come ad esempio l'introduzione dell'agente provocatore. Checché ne dica il senatore Caliendo - riprendo alcune parole che aveva detto - qui c'è una vera e propria epidemia di corruzione. Siamo di fronte ad un'epidemia, che non si cura con l'aspirina, ma con l'accetta

dei soldi che arrivano da «qualcosa» e mi compro una casa per uso personale, non è autoriciclaggio. È una norma quantomeno singolare; forse bisognava intervenire su quanto approvato. Perché non si può intervenire su una misura introdotta da poco da questa maggioranza e da questo Governo facendola diventare una cosa seria?

il popolo, neanche noi possiamo accettare compromessi al ribasso, perché questo è quello che fanno gli altri: accettano compromessi al ribasso. Ma il compromesso, se è una parola che avrebbe un senso e potrebbe essere importante, o è alto o non è altrimenti non usciremo mai vivi da qua dentro. Non usciremo vivi e non faremo mai veramente gli interessi della gente se non iniziamo a capire che la parola compromesso

Vogliamo arrivare a fare una cosa veramente seria? Eliminiamo il compromesso al ribasso e andiamo verso un compromesso al rialzo, alto, forte, altrimenti non ha senso il nostro e il vostro stare qua dentro. Noi ci apprestiamo a esprimere questo voto con le spalle forti, di chi ha chiesto alla propria gente, anzi ai cittadini che liberamente si sono iscritti al nostro portale, cosa ne pensano. Abbiamo chiesto a loro, e loro ci hanno detto di votare no, e sono coloro che noi siamo qui dentro a rappresentare. Siamo in una democrazia rappresentativa? Rappresentiamo i cittadini? Chiediamo un po' ai cittadini cosa ne pensano. Questo dobbiamo fare. Se chiedete ai cittadini, i cittadini studiano molto più di quello che noi pensiamo, perché noi non siamo quello che una volta si chiamava *intellighenzia*. No, per piacere, no. I cittadini devono studiare e, studiando, si informano ed esprimono coscienziosamente il loro pensiero. Non pensiamo di essere al di sopra dei cittadini, altrimenti siamo finiti. Per fare una buona legge anticorruzione non è sufficiente il titolo. Le parole di Pertini sono molto chiare e quanto mai attuali; quindi, il nostro voto non potrà che essere contrario, però, veramente, vi spingo ad amare voi stessi: amate voi stessi e amate il popolo che dite di rappresentare. Ogni tanto facciamo qualcosa nel pieno e concreto interesse. Non possiamo accontentarci di una mezza cosa. Una cosa sana la riuscirete mai a fare?

Signor Presidente, signor Ministro, signori del Governo, colleghi,

i rapporti commerciali tra imprese, alterando la *par condicio* ed incidendo negativamente sulla libera concorrenza.

La sanzione penale è l'*extrema ratio*; la nostra democrazia si fonda sul corretto funzionamento del sistema dei controlli (controlli in via amministrativa, controlli che riguardano le istituzioni). Signor Ministro, il nostro no è anche una scommessa,

Io sono abituato a dire sempre quello che penso, per cui non accetto chi fa lezioni moralistiche

quando Forza Italia non ha preteso di andare alle elezioni e si è formato un Governo tecnico, nonostante Berlusconi avesse avuto già una prima condanna. È facile dunque fare il moralista oggi. Vorrei

Lei sa benissimo che abbiamo dovuto presentare gli emendamenti il giorno prima che la Camera approvasse la riforma della prescrizione,

Senatore Lumia, se mi distrae il Ministro non riesco a fargli capire qual è la nostra speranza,

Quando ci troviamo di fronte a pene che non corrispondono più a quello che è l'impianto dell'equilibrio del sistema sanzionatorio, non vi è

vanno tenuti fuori tutti coloro che vengono intercettati e che non c'entrano con i delitti. Con queste norme avete invece aumentato a dismisura

la lotta al terrorismo e alla mafia in questo Paese l'abbiamo fatta senza intercettazioni e senza norme speciali. Falcone ha fatto il grande processo alla mafia seguendo il percorso del denaro e non con le intercettazioni. Queste erano le regole,

Noi rispondevamo che ciò era sbagliato, perché la sanzione penale deve riguardare solo pochi fatti e, per essere effettiva, deve essere irrogata in poco tempo.

Come posso votare una legge che, oltre a tradire sotto questo aspetto i principi costituzionali, introduce alcuni aspetti veramente contrari

accertare la responsabilità e non creare la norma, non deve essere l'arbitro del lecito e dell'illecito, individuando qual è l'illecito

sulla riduzione del minimo della pena, lasciando a lei la responsabilità politica di riequilibrare i massimi di pena con i termini di prescrizione. Sul falso in bilancio avevamo proposto pochi emendamenti, che servivano però a rendere costituzionale quella norma, che invece non solo è incostituzionale perché lascia al giudice

come fossero qualcosa che è al di fuori, dicendo che sono importanti: anche dire ciò significa stabilire un limite tra i fatti materiali rilevanti e quelli di lieve entità. Da ultimo,

al povero Cristo, a cui viene sottratta la pensione, o all'evasore fiscale, che non restituisce nulla allo Stato. Noi non abbiamo detto che la norma non va bene, abbiamo detto: rendiamola costituzionale, quindi che valga sia per i corrotti che per gli autori di altri reati. E vado alla conclusione. Se questi sono i principi costituzionali, mi domando, signor Ministro, per quale motivo si sia scelta la strada di non trovare un accordo. Eppure, il suo emendamento sulla materia del falso in bilancio conteneva giustamente tutti gli elementi per una corretta azione di contrasto alla corruzione. Ed invece l'ha cambiato, con un ulteriore emendamento.

pensano che attraverso l'aumento della pena si sono messi la coscienza a posto. L'aumento di pena l'avevamo già introdotto nel 2012, ma non è venuto meno nulla.

avranno dato miglior risultati o addirittura avranno aggravato la situazione della corruzione nel nostro Paese. Per queste ragioni, il Gruppo

il senatore Schifani ha ben esposto il contenuto di gran parte del provvedimento, di cui quindi ricorderò soltanto due norme: l'allungamento dei tempi della prescrizione e la reintroduzione del falso in bilancio. Sono norme che erano già presenti nel nostro ordinamento e che nel recente passato furono modificate o soppresse, con effetti molto negativi per la giustizia. Adesso stiamo ripristinandole. Qualcuno ha sostenuto che prescrizione e falso in bilancio non avrebbero alcun rapporto con la corruzione, mentre è vero esattamente il contrario. La prescrizione corta spesso non consente di punire i corruttori ed i corrotti, che oggi operano con tecniche e mezzi molto sofisticati, con triangolazioni così sottili e mimetizzate da rendere necessarie indagini molto lunghe e complesse. Considerazioni analoghe valgono per il falso in bilancio, previsto pressoché in tutti gli Stati di diritto. La falsificazione del bilancio, oltre a rendere opaco il mercato, è anche il mezzo tecnico usato per costituire i fondi neri, neri, necessari per alimentare la corruzione. Non stiamo parlando tanto dell'errore materiale del ragioniere che prepara il bilancio di una piccola società, quanto dell'artificio doloso che nelle imprese serve a costituire un tesoretto occulto, pronto per mille usi. E diciamolo chiaro: senza fondi neri la corruzione diventa molto difficile e spesso impossibile. Sarebbero sufficienti queste due norme per aprire uno spiraglio di luce nella durissima guerra contro la corruzione e per meritare il voto anche di chi, come il Movimento 5 Stelle, poco fa ha dichiarato che farà diversamente, pur avendo concordato in Commissione numerosi e decisivi punti del provvedimento. Capisco questo metodo di affidarsi ai sondaggi, ma debbo ricordare ai colleghi del Movimento 5 Stelle che il Parlamento è cosa diversa dai loro sondaggi. *(Applausi Ma c'è altro da aggiungere. La rigenerazione dell'Autorità anticorruzione e l'indirizzo serio e concreto che le ha dato il presidente Cantone.

Presidente, posso continuare? L'approvazione del reato di autoriciclaggio che punisce i sotterfugi volti a rendere irriconoscibile l'utilizzo delle risorse provenienti dalla corruzione.

che sana una grave lacuna della nostra legislazione penale. Sono tutte norme attese da molti lustri, che indicano con chiarezza la politica del Parlamento e del Governo. Ciò nonostante, l'umore e il sentimento di fondo emersi nel nostro dibattito segnalano che tutto il lavoro fatto nell'ultimo anno, pur positivo, per quanto necessario, non è ancora sufficiente. Sappiamo che in Italia la corruzione e la collusione, per dimensioni, radicamento e modalità di esercizio, hanno assunto la forma di un'idra a mille teste, che più si tagliano, più ricrescono. Ogni giorno apprendiamo con vergogna l'esito di nuove inchieste, che toccano tutti i rami della vita economica, sociale e politica del Paese, coinvolgono imprese, pubblica amministrazione e politica, compresi esponenti del mio partito. La corruzione arriva anche a lambire uomini delle Forze dell'ordine, della magistratura e della Chiesa. Davanti a un inquinamento così profondo e capillare, il Parlamento non può non sapere che le buone leggi non bastano, che per battere la corruzione bisogna arrivare al cuore della malattia e comprendere le cause e le ragioni che hanno reso possibile una pratica così vasta. Accanto alla crisi morale che tocca tanta parte della società, c'è il progressivo, profondo indebolimento dello Stato. Negli ultimi decenni, il nostro Stato si è infragilito in tutte le sue principali articolazioni, dai poteri costituzionali ai grandi servizi pubblici, dal reticolo delle autonomie all'insieme della pubblica amministrazione. Senza uno Stato che funzioni sulla base di regole chiare, che garantisca il rispetto delle procedure, che verifichi, controlli e sanzioni, il minimo che può succedere è l'espandersi della corruzione, dalla criminalità, dell'evasione e dell'elusione fiscale. Oggi dobbiamo dire che per sradicare la corruzione, oltre all'azione della giustizia, serve l'impegno quotidiano di tutte le forze dello Stato; serve un ambiente pubblico che non la faciliti ma, al contrario, la contrasti levandole l'acqua in cui sguazza. Se le forze dello Stato non operano in un solido spirito di legalità, è molto difficile che questo spirito possa essere trasmesso ai cittadini e alle forze economiche. della realizzazione delle grandi opere pubbliche è stata affidata all'ingegner Incalza nel 2001 dal ministro Lunardi. Non rileva, in questa sede, che già allora Incalza fosse stato coinvolto in vicende giudiziarie; rileva, invece, che, salvo la breve parentesi del ministro Di Pietro, Incalza abbia mantenuto ininterrottamente quella responsabilità sino a poche settimane fa, e cioè per ben quindici anni. Questo è il nodo è il nodo politico. La corruzione e la collusione si vincono in primo luogo con la vigilanza, il controllo, l'azione preventiva della pubblica amministrazione e dei suoi corpi tecnici. Nei primi decenni del dopoguerra, la ricostruzione e la modernizzazione del nostro Paese sono state possibili anche per il contributo e l'alta professionalità di tanti uffici del genio civile e dell'ANAS, per l'illuminato avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Dobbiamo chiederci perché tanto patrimonio tecnico sia andato dissolvendosi. Se, per inettitudine o dolo, il primo ed essenziale baluardo contro la corruzione, quello della pubblica amministrazione, viene a mancare, la battaglia è già persa. La magistratura, anche la più severa ed efficiente, non sarà mai in grado di farcela da sola. A un mandato di impropria lunghezza come quello di Incalza, avrebbe dovuto corrispondere il controllo, passo dopo passo, dell'autorità politica. Considerazioni analoghe possiamo fare sugli effetti disastrosi della legge obiettivo. Voluta nel 2001 per sveltire i grandi lavori pubblici, in quattordici anni ha completato solo l'8 per cento delle opere programmate e ha registrato un aumento dei costi del 40 È dal 2003 che vengono denunciati, senza alcun esito, i drammatici effetti di una legge che fa dell'impresa costruttrice il *dominus* anche della progettazione e della direzione lavori. È questa incredibile concentrazione di poteri in capo a un soggetto portatore di propri interessi economici a costituire terreno propizio per ogni degenerazione. Come si può pensare che, con leggi simili, i progetti non vengano piegati all'interesse imprenditoriale ed economico dell'impresa e i controlli non vengano addomesticati con gli stessi fini? Leggi sbagliate, messe a disposizione di mani fameliche non possono non produrre effetti gravemente Oggi l'Italia mostra di voler risalire la china. Le previsioni sul PIL sono passate dal segno meno al segno più: è un segnale piccolo, ma dobbiamo coglierlo. Il prezzo del petrolio, il rapporto dollaro-euro, lo *spread* ridotto sono tutti fattori che debbono spingerci a fare di più e a cogliere opportunità che non si manifestavano da almeno sette anni. In questo scenario la lotta alla corruzione e all'evasione fiscale debbono costituire una priorità nazionale assoluta. Battere la corruzione è in primo luogo un imperativo etico, ma è anche una condizione essenziale per favorire la ripresa, attirare investimenti, ridare forza al mercato. L'impegno dei senatori del Partito Democratico non si esaurirà con l'approvazione del disegno di legge in esame, con il voto di questo pomeriggio: sappiamo che è molto utile, ma sappiamo anche che non è sufficiente. Noi vogliamo contribuire a fare chiarezza e trasparenza su una fase così difficile della nostra storia e lo facciamo con due impegni politici precisi. In primo il Partito Democratico in Senato assume come priorità assoluta l'approvazione del nuovo codice degli appalti, che oggi è all'esame della Commissione, e indica sin d'ora la propria volontà a farne non solo uno strumento utile allo sviluppo della nostra economia, ma anche un passo essenziale per battere ogni corruzione. L'obiettivo è arrivare a un assetto efficiente della legislazione dei contratti pubblici e al rafforzamento delle autorità e delle istituzioni preposte al controllo e alla tutela della concorrenza nelle commesse pubbliche. In secondo nei mesi passati i senatori del Partito Democratico hanno presentato un disegno di legge per la costituzione di una Commissione d'inchiesta sull'ANAS, ma i risultati delle inchieste che stanno emergendo inducono ad ampliare l'iniziativa. Nei prossimi giorni proporremo, quindi, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione. II Parlamento deve stare molto attento a non sovrapporsi al lavoro della magistratura, ma ha il dovere di valutare i fatti corruttivi assieme alle loro interconnessioni con l'economia, le imprese, la finanza, la criminalità - anche internazionale -, la politica, le istituzioni e la pubblica amministrazione. Il bubbone corruttivo è così complesso e intrecciato con i fatti della vita politica, economica e sociale del Paese da obbligarci a un'analisi di verità e a tutte le conseguenti assunzioni di responsabilità della politica. Ce ne occuperemo con lo strumento più incisivo che la Costituzione e i nostri Regolamenti ci mettono a disposizione. Prima di passare alla votazione finale, avverto che il relatore ha presentato una proposta di coordinamento che è in distribuzione. Chiedo al relatore, senatore D'ascola, se intende illustrarla. si tratta di una illustrazione estremamente limitata. Noi abbiamo approvato l'emendamento 6.300, a firma del senatore Lo Giudice, il quale introduce tutta una serie di disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena con riferimento all'articolo 165 del codice penale. Data quindi la specificità della questione modificativa, integrativa - per meglio dire - del testo dell'articolo 165, il relatore si permette di ritenere che forse questo emendamento dovrebbe trovare un'allocazione specifica in un articolo autonomo di questa legge.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente. Nella seduta di oggi, a conclusione del disegno di legge sulla corruzione, si procederà allo svolgimento delle relazioni sul collegato in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e sul disegno di legge concernente misure cautelari personali. La seduta di domani sarà limitata alla trattazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Matteoli. I lavori della prossima settimana riprenderanno alle ore 11 di mercoledì 8 aprile, con il seguito della discussione del disegno di legge collegato sulle amministrazioni pubbliche. Per tale provvedimento, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 13 dello stesso giorno. Il calendario prevede quindi l'esame di ratifiche di accordi internazionali, il seguito del disegno di legge recante misure cautelari personali, l'esame del disegno di legge collegato in materia di agricoltura e, a seguire, gli altri argomenti già indicati. **Calendario dei

considerato che il collegato è stato ampiamente modificato durante i lavori in Commissione. Se fosse stato approvato nella sua forma originale, gli emendamenti potevano essere ripresentati così com'erano, trattandosi di un collegato.

mi preme dire che la richiesta del presidente Crimi ha ad oggetto un provvedimento molto complesso e profondamente cambiato dalla Commissione, tanto che gli emendamenti presentati in quella sede, anche mantenendo lo stesso identico oggetto, devono essere riferiti ad un diverso testo.

ha esitato, con i suoi pareri, la vita o la morte di alcuni emendamenti. Penso, pertanto, che sia diritto dei Gruppi parlamentari poter rivedere, anche alla luce dei pareri della Commissione bilancio,

Onorevoli colleghi, in relazione al procedimento avviato su denuncia di alcuni senatori dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma sui sui fatti accaduti nella seduta pomeridiana del 5 novembre 2014 nell'Aula del Senato, nell'ambito del quale sono stati chiamati a testimoniare alcuni senatori, tra cui due senatori Questori, ho ritenuto, acquisito l'avviso unanime dei Capigruppo, dei Vice Presidenti e dei senatori Questori, di scrivere al procuratore della Repubblica per affermare il difetto assoluto di giurisdizione della magistratura ordinaria

ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996, secondo la quale l'attività posta in essere dai membri delle Camere non può formare oggetto di attività inquisitiva del pubblico ministero né di accertamento da parte del giudice. Ho chiesto pertanto alla procura che il procedimento e la convocazione di testimoni non abbiano ulteriore seguito. Della questione sarà altresì investita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per le valutazioni di competenza. Tanto era dovuto secondo le decisioni della riunione.

Consentite al senatore Pagliari di svolgere il suo intervento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo periodo mi sono sentito ripetere più volte: riforma della pubblica amministrazione? Non penserà il *Premier* di riuscire in quello in cui non sono riusciti illustri Presidenti e Ministri del calibro di Massimo Severo Giannini? È uno sforzo inutile.

Vero è il riferimento storico, e legittimo il pessimismo della ragione. L'ottimismo della volontà però è un dovere imprescindibile per la politica, per il Parlamento e per il Governo. La responsabilità della politica è di dare soluzione ai problemi veri, di non arrendersi e di scegliere non in modo tattico ma in chiave strategica, mettendoci la faccia, proponendo soluzioni vere, anche se difficili e scomode, altrimenti lo sforzo sarebbe inutile e di facciata. Tutto questo presuppone che vi sia una vera necessità da soddisfare, una questione reale. perché la riforma della pubblica amministrazione? Tutto oggi dice, con evidenza assoluta, che per la pubblica amministrazione non basta voltar pagina ma è necessario cambiare libro. Perché? Per la corruzione? Certamente. Ma non solo. E vorrei dire non prioritariamente. C'è una pubblica amministrazione vissuta come ostacolo, c'è una legalità vista come un inutile orpello, ci sono imprese e privati che restano senza risposte e subiscono inutili ritardi e freni nelle loro attività. Tutto questo evidenzia lo iato tra la Costituzione materiale e la Costituzione formale, articoli 97 e 98 della Costituzione, che postulano il buon andamento, l'imparzialità e il servizio esclusivo della Nazione. infatti, è troppo spesso, anche nell'ottica del valore costituzionale della leale collaborazione, un corpo a sé, un tendenziale contropotere portato ad andare oltre, mentre deve essere un potere che resta nel suo ambito. Questo dato, senza fare di ogni erba un fascio, mi sembra purtroppo innegabile. Quali le cause? Tante: debolezza della politica, *deficit* tecnico del sistema, logica del contropotere, crisi del sistema, inefficacia dei controlli, rapporti innaturali tra politica e amministrazione, responsabilità come *optional*, legislazione elefantiaca, disarmanti lentezze della giustizia. Sotto questo profilo, sarebbe lunga la riflessione sull'inadeguata applicazione della divisione tra tecnica e politica, con la prevaricazione dei politici sui tecnici con scarsa dignità e professionalità e dei tecnici sui politici con pari scarsa dignità e professionalità. Ma c'è più in generale un tema, quello dei tecnici che agiscono guidati dal principio della transitorietà dei politici. I recentissimi scandali ne sono un emblematico e poliforme esempio. Il punto è dunque quello una volta ancora con l'ottimismo della volontà, un processo di ricostruzione e di rimodellazione della pubblica amministrazione, nell'ottica degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Si tratta di un processo che comporta un cambio di contesto ordinamentale non meno di un cambio di costume e di mentalità e che chiede alla politica il coraggio di promuovere questo cambiamento. Ebbene, sia per l'impianto originale del decreto-legge di iniziativa del ministro Madia, sia per lo sforzo compiuto da voi colleghi con gli emendamenti, dalla Commissione affari costituzionali e - se permesso - da me come relatore, in un dialogo costruttivo e fattivo con il Ministro stesso e con il suo pregevolissimo *staff*, nella proposta che viene presentata alla nostra attenzione ci sono scelte che potenzialmente vanno nel senso giusto. cittadinanza digitale cerca di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale con misure molteplici, delle quali a mio parere meritano particolare menzione quelle sull'abbattimento delle barriere concrete di accesso e di rapporto tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini e quelle sull'educazione informatica di questi ultimi, che è un elemento di democrazia nell'evoluzione della nostra società. Gli articoli 2 e 3 riguardano la disciplina dell'attività amministrativa, uno dei profili cardine di una riforma della pubblica amministrazione. La legalità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione dipendono dalla puntualità, tempestività ed esatta modulazione della decisioni. Queste disposizioni si incentrano soprattutto sui meccanismi procedimentali, garantendo l'esercizio delle funzioni di ogni amministrazione coinvolta in tempi tali che non consentano l'eternalizzazione di fatto dei procedimenti e delle decisioni; una eternalizzazione che rende "schiavo" il privato e rende "schiava" l'impresa che attende risposte dalla pubblica amministrazione. In questa chiave si muovono le proposte, contenute nell'articolo 2, su quell'istituto fondamentale che è la Conferenza dei servizi. In questa disciplina si introducono elementi che garantiscono una decisione certa e in tempi predefiniti, che portano che portano il rapporto all'interno della Conferenza dei servizi nell'ottica della leale collaborazione fra amministrazioni e che quindi consentono di valorizzare questo strumento. Così è per il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche,

ma non impedendo la conclusione dei procedimenti che sono nell'interesse dei cittadini e delle imprese. Sempre alle attività si riferisce l'articolo 4, che io credo sia una norma fondamentale perché, attraverso l'esercizio della delega ivi questo Paese avrà finalmente la disciplina delle attività assoggettate, nelle diverse forme, ad una semplice comunicazione del privato e delle imprese. Il nostro ordinamento si è andato evolvendo da un ordinamento dell'autorizzazione preventiva ad un ordinamento del controllo successivo, da un'amministrazione autorizzativa ad un'amministrazione del consenso. Questa trasformazione, che è avvenuta di fatto nella legislazione, non ha mai trovato punti di definizione e di regolazione organica, e questa è la prima occasione perché, attraverso questa delega, dando una disciplina concreta a queste attività di iniziativa dei privati, si realizza un contesto di garanzia e di certezza giuridica dei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione. Si creano condizioni per le quali queste attività, che iniziano per opera del privato, e che trovano nell'amministrazione solo la possibilità del controllo, possono svilupparsi in questa logica, senza che intervengano quei fenomeni distorsivi che il timore di perdita di potere da parte della burocrazia ci ha portato a verificare, giorno dopo giorno, nella realtà dei Comuni e delle amministrazioni pubbliche. Dare certezza su questo vuol dire dare un profondo contributo a quella ridefinizione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, che deve andare nel senso di un'amministrazione che, garantendo la legalità, non è contro il cittadino, ma è nella logica dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, della solidarietà e cioè è strumento dell'affermazione e dello sviluppo dell'iniziativa del privato. Non meno significativo sul piano della certezza dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini è l'articolo 5, con la nuova disciplina questo è un elemento tecnico - per esempio, dell'annullamento d'ufficio, con l'individuazione di un termine certo entro il quale questo annullamento può essere esercitato (che sono i 18 mesi). Ricordo anche l'articolo 6, la delega sul diritto all'accesso dei parlamentari, che porrà fine a prassi incostituzionali, e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciute ai gestori delle reti telefoniche per le intercettazioni e le altre attività attività d'indagine; un contributo forte, anche questo, nel senso del processo della lotta alla corruzione. Gli articoli 7 e seguenti spostano l'attenzione sui profili organizzativi Nell'articolo 7 si prevede la riduzione degli apparati strumentali, il riordino e la razionalizzazione delle funzioni di polizia; il riordino delle funzioni di tutela dell'ambiente, del territorio, del mare, dei controlli nel settore agroalimentare, con la riorganizzazione del corpo forestale dello Stato e il suo eventuale accorpamento; un riordino delle funzioni della Presidenza del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 95, del suo potere di indirizzo e della responsabilità della collegialità dell'azione del Governo. C'è la previsione relativa agli uffici territoriali periferici dello Stato, una misura molto importante e molto significativa non solo perché dà sul territorio un coordinamento alla presenza dello Stato, ma anche perché, attraverso questa riorganizzazione, che sarà anche di tipo logistico, si avrà la possibilità, anche nell'ottica della Conferenza dei servizi, di avere una rappresentanza unitaria sul territorio, e in periferia delle rappresentanze dello Stato. E chi chi opera nella pratica delle amministrazioni sa quanto ciò sia importante e quanto possa aiutare a definire e a restringere i tempi di decisione e a chiarire i rapporti di collaborazione e di interazione tra privati e imprese e pubblica amministrazione.

vista la censura fatta dalla Commissione bilancio sull'articolo 9. Si tratta di una ridefinizione delle Camere di commercio che, comportando una riorganizzazione dal punto di vista numerico, mantenendo il registro delle imprese e con una riorganizzazione e una ridefinizione dello stesso assetto delle partecipazioni delle Camere di commercio,

una misura di certo rinnovamento del sistema delle Camere di commercio: sono misure che non credo nessuno possa prendere come punitive o come antitetiche o oppositive. Sono misure che vanno nel segno di di quel processo di modernizzazione che, senza retorica, tutti avvertiamo che dovrebbe essere proprio delle pubbliche amministrazioni. In questa stessa logica

Tutti sappiamo qual è l'importanza anche economica dei servizi pubblici locali; tutti sappiamo qual è l'importanza del settore della società partecipate e quale quale potenzialità questo settore può avere per l'azione dei pubblici poteri, ma anche quanto esso abbia contribuito, purtroppo negativamente, diventando

innanzitutto, la riduzione del numero delle società partecipate; il collegamento alle funzioni istituzionali delle amministrazioni partecipanti;

quella che penso sia una misura assolutamente importante, introdotta dal Parlamento, vale a dire una disciplina della responsabilità che prevede la responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti. Ciò vuol dire che nelle società partecipate

amministratori pubblici andavano ad imporre le scelte, spostando il debito sulle società partecipate, così facendo clientela a livello di assunzioni e a livello di consulenze in queste stesse società. Attuare questa delega vuol dire realizzare un'importante inversione di tendenza sulla prassi e sull'uso di meccanismi che hanno una loro potenzialità, ma vuol dire anche incidere su comportamenti e costumi politici, proprio nella logica di quello che è stato deciso poco prima dell'anticorruzione. Non meno importante è l'articolo 15, sui servizi pubblici locali, in cui si ribadisce la funzione fondamentale che questi servizi svolgono e la loro finalizzazione alla soddisfazione dei bisogni della collettività in una chiara chiave di aggancio con l'uguaglianza sostanziale dell'articolo 3, in cui è prevista una disciplina

aggregazioni, oltre a regimi tariffari che prevedano che gli eventuali incrementi di produttività vengano destinati a ridurre l'aggravio dei servizi su imprese e cittadini. Torno adesso sull'altro tema che sull'altro tema che attiene sempre alla riorganizzazione: mi riferisco al tema dei dipendenti pubblici. Ci sono due norme che riguardano questo aspetto: l'articolo 13 sul Testo unico sul lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e l'articolo 10. Questi due articoli sono legati tra loro da un filo: è il filo che parte dalla considerazione che il luogo comune dei dipendenti pubblici fannulloni è, appunto, un luogo comune e che c'è una valorizzazione del personale pubblico da fare. una valorizzazione che non deve fare di ogni erba un fascio, né in positivo, né in negativo, e che, quindi, deve impedire che i bravi dipendenti pubblici vengano accusati di essere fannulloni, ma che non deve impedire che i fannulloni nella pubblica amministrazione portino il peso e le conseguenze del mancato adempimento delle loro funzioni. In questa chiave, ci sono delle norme generali, cioè quelle dell'articolo 13 del Testo unico, che vanno nel senso del miglioramento del miglioramento della qualità delle condizioni di espletamento dei concorsi che vengono accentrati e della ricerca di metodi di selezione che siano più adeguati alla ricerca delle professionalità e, quindi, alla valorizzazione dei cervelli, più che alla valorizzazione delle conoscenze puramente delle conoscenze puramente nozionistiche che vanno ad accentuare il tema della valutazione del merito dei dipendenti pubblici rispetto alle valutazioni formali che caratterizzano il sistema attuale. C'è poi l'articolo 10 sulla sulla dirigenza pubblica, che è sicuramente uno degli articoli che maggiormente ha accentrato l'attenzione dell'opinione pubblica. Da questo punto di vista, vorrei subito dire che il tema non è quello dei segretari comunali. Il tema dei segretari comunali lo abbiamo risolto

dovevano essere oggetto di riforma. Questa è però una riforma che colpisce, perché, nella logica di superare la crisi della pubblica amministrazione, si permette di pensare ad una dirigenza che muti completamente le sue le sue condizioni, le sue radici, il contesto di operatività: non condizioni che vengono mutate per togliere garanzie, ma condizioni che vengono mutate per valorizzare la funzione e l'importanza della dirigenza; per consentire che la dirigenza possa esprimersi al meglio nella distinzione tra tecnica e politica e possa dare il suo contributo imprescindibile. Per questo non abbiamo però bisogno di burocrati che si consolidano in un posto e in quel posto rimangono, di burocrati che conoscono semplicemente una fetta e su quella fetta costruiscono la loro fortuna personale e magari anche la loro fetta di potere. Abbiamo bisogno di una dirigenza che, proprio perché professionale, sappia che il principio del concorso sul piano professionale, della necessità del costante aggiornamento, della necessità di mettersi sempre in discussione è il qualcosa che serve. Infatti, abbiamo bisogno di una dirigenza che possa rendere dinamica la nostra pubblica amministrazione e questa dirigenza è solo quella che sa di essere messa continuamente in discussione sul piano professionale, di doversi riguadagnare, tempo dopo tempo, la funzione, la collocazione ed il prestigio del ruolo e di doversi confrontare senza limiti

delle correnti interne alle amministrazioni. È una sfida alla dignità e alla professionalità vera: quella professionalità che si gioca sulla capacità di esercitare le proprie funzioni tecniche e di esercitarle nel contesto di una deontologia vera. C'è poi l'articolo 15*-bis*, che si collega a questo tema appena toccato. L'articolo 15*-bis* è quello che introduce una delega che consentirà eliminare entro 90 giorni tutte quelle previsioni di decreti ministeriali e di regolamenti attuativi che hanno impedito l'entrata in vigore di tante normative. Sappiamo dalla prassi che questi decreti ministeriali e questi regolamenti attuativi sono stati spesso, nell'uso distorto e nella strumentalizzazione di tali previsioni, lo strumento per impedire che leggi non gradite entrassero in vigore. Anche questa è una misura di forte e significativa di forte e significativa incidenza su processi che bloccano il corretto rapporto tra il potere legislativo, il potere esecutivo e l'amministrazione tutta.

del sistema dei controlli, di una ridefinizione del processo contabile e di aggredire il tema della semplificazione normativa. Non possiamo più pensare che, nell'ambito della riforma complessiva dello Stato italiano, non ci sia e non ci debba essere l'individuazione di un modo di legiferare, che dia ordine, certezza e conoscibilità immediata ai testi e alle loro modifiche.

non sarà possibile se non ci sarà una riforma e un efficientamento complessivi del nostro sistema pubblico. Questo efficientamento complessivo, a mio modo di vedere, non può non partire da un efficientamento vero e deciso del sistema giudiziario italiano *(Applausi del senatore Cuomo)* sia esso civile, penale, amministrativo, tributario o contabile. Tutte le riforme della giustizia saranno senza futuro, sino a quando non partiremo dalla regola essenziale di fissare tempi certi, nella flessibilità intelligente della norma, per la definizione del giudizio. un tempo certo per l'azione della pubblica amministrazione: perché non ci deve essere un tempo certo per l'azione giudiziaria? Ciò non incide né sull'indipendenza, né sull'autonomia, né sullo svolgimento della funzione, ma fa assumere a carico anche del sistema giudiziario - quindi degli avvocati, così come dei magistrati - il problema di non negare giustizia e di dare quindi una risposta vera, forte ed efficace.

Ho notato una grande resistenza al cambiamento e una difficoltà a capire che il cambiamento è interesse di tutti.

del cambiamento, che dobbiamo accettare di metterci in discussione, non per fare piacere a questo o ad un altro Presidente del Consiglio, ma perché si tratta di un problema che, se lo vogliamo

insieme, non riusciremo a sviluppare tutte queste potenzialità. Voglio ringraziare il Ministro per la collaborazione. Abbiamo collaborato in un confronto molto aperto e dialettico, ma sempre profondamente costruttivo. Credo che il Parlamento giudicherà i risultati di questo confronto ma, con la consapevolezza dei limiti, credo che un certo lavoro sia stato svolto. Voglio ringraziare la Presidente della Commissione affari costituzionali, cui devo l'opportunità di questa esperienza, senatrice Lo Moro, e tutti i componenti della Commissione affari costituzionali e non me ne vorranno quelli degli altri partiti se prima di tutto ringrazierò i miei colleghi di partito, che mi sono stati amici e dei quali ho sentito il sostegno in tutto il percorso.

mi limiterò ad alcuni riferimenti rispetto ad un testo legislativo estremamente complesso, il volto del quale, ciononostante, credo di poter sufficientemente dettagliare

Intanto, dal riferimento all'attualità delle esigenze cautelari, una ulteriore circostanza che è volta a rendere ancora più dettagliata e specifica la motivazione. Vedremo poi quali altre disposizioni si riflettono sulla struttura della motivazione, che deve essere data a giustificazione della limitazione della libertà personale come anche di quelle libertà sacrificate da misure di natura interdittiva. C'è poi un ulteriore riferimento che, in un certo senso, risolve una questione giurisprudenziale estremamente nota, allorquando si dice che le esigenze cautelari, oltre che attuali, non possono essere desunte dalla gravità del titolo del reato. la valutazione deve essere sempre pertinente, specifica e riferirsi al caso concreto e non di tipo generalizzante, cosa che comporterebbe di escludere, ovviamente per reati molto gravi, la possibilità che l'imputato venga perseguito, come una volta si diceva con espressione diffusa all'interno dei tribunali, a piede libero. La La possibilità di emissione di misure coercitive non è quindi condizionata dalla gravità: anche per un reato estremamente grave l'imputato potrà trovarsi in stato di libertà personale ovviamente il piano determinativo della restrizione della sua libertà personale sarà determinato, per un verso, dalla gravità degli elementi indiziari, per altro verso, da un panorama di esigenze cautelari effettivamente giustificativo della restrizione della libertà personale, come anche delle altre libertà connesse alla applicazione di eventuali misure interdittive. estremamente interessante, se mi è consentito soffermarmi, sempre brevemente, su questo tema, è quello connesso all'articolo 275,

È nota la circostanza di una legislazione frequentemente modificata, non soltanto dagli interventi legislativi, ma anche da quelli della Corte costituzionale,

del 2015 (udienza del 25 febbraio, se la memoria non mi inganna), con la quale la Corte costituzionale, interpretando un riferimento al 416-*bis* del codice penale, ha ritenuto di escludere il concorso esterno

rispetto al passato. Abbiamo i tre reati ai quali ho fatto riferimento e per i quali si afferma la presunzione di esigenze cautelari, sia pure con quella espressione che la relativizza: «salvo che siano acquisiti esigenze cautelari». C'è poi una seconda categoria di reati, quelli di cui ad esempio all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, ossia le norme che dettano disposizioni organizzative degli uffici distrettuali

più drastici, inevitabilmente nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla giurisprudenza costituzionale, in virtù delle quali si dice, ulteriormente, che non soltanto si deve valutare se non esistano ragioni che escludano la sussistenza delle esigenze cautelari, ma si deve anche valutare se per caso quelle esigenze cautelari possano anche essere anche neutralizzate dall'adozione di provvedimenti diversi rispetto a quelli concernenti l'instaurazione della custodia cautelare in carcere. Quanto alla struttura della motivazione - ne parlavo per l'appunto poc'anzi - si introduce una componente di motivazione: si deve spiegare il perché

la misura degli arresti domiciliari sostanzialmente centrale dal punto di vista della possibilità di instaurazione di una misura cautelare limitativa della libertà personale, dal momento che si deve preliminarmente spiegare per quale ragione dovrebbero risultare insufficienti gli arresti domiciliari e, di conseguenza, sul piano interpretativo - credo che non sia possibile giungere a diversa conclusione - la custodia cautelare in carcere rappresenta una soluzione residuale perché da adottarsi tutte le volte in cui si deve spiegare che gli arresti domiciliari costituirebbero un provvedimento inefficace sul necessario versante della neutralizzazione delle esigenze cautelari. poi disposizioni dettate per il caso di trasgressione delle cautele connesse, ad esempio, ad una misura cautelare degli arresti domiciliari. La possibilità, legata soltanto a fatti di lieve entità, di nuova concessione di arresti domiciliari a soggetti condannati per evasione, è possibile soltanto per evasione nel quinquennio, ed è possibile soltanto allorquando la trasgressione venga ritenuta dal

deve implicare una necessaria autonomia nella valutazione delle singole specifiche esigenze cautelari, perché poi la mancata valutazione autonoma delle singole esigenze cautelari determinerebbe anche un vizio di motivazione - è scritto

questa professione e questa attività l'hanno svolta, a prescindere dall'essere magistrati o avvocati - che il problema dell'autonomia, ossia della necessità di dettare un autonomo segmento all'interno della motivazione per le esigenze cautelari che vengono rappresentate, abbia costituito oggetto di dibattito, ma anche di opportuni interventi della Corte Corte di cassazione. In fondo, in questo caso non si fa altro che prendere parti del dibattito giurisprudenziale sul punto e renderle - per l'appunto - norma. Si dispone, anche in questo caso prendendo atto di alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione, la necessità della comparizione dell'imputato in occasione della camera di consiglio che si celebra davanti al Tribunale della libertà. Sappiamo che è un'interpretazione (che la Corte di cassazione aveva

se compare (quindi con quel «se» che rendeva la comparizione una vera e propria eccezione), aveva determinato taluni arresti giurisprudenziali, soprattutto di merito, a ritenere la presenza dell'imputato del tutto facoltativa. che questa sia una scelta garantista, di libertà: insomma, se è in discussione la libertà personale e se quel soggetto può contribuire a chiarire dinanzi al giudice del processo endoprocessuale la sua posizione, lo deve fare non attraverso il giudice di sorveglianza, che trasmetterebbe un verbale privo della pregnanza della diretta comunicazione che si connette a un vero e proprio interrogatorio: deve poter comunicare le ragioni della sua difesa.

dalla difesa materiale, che compete ovviamente all'imputato: lui sa cosa poter dire e cosa conosce dei fatti; chiaramente, il difensore non può mai costituire un tramite, anche perché frequentemente è all'oscuro della realtà dei fatti, ma non può certamente costituire un tramite della difesa materiale da riconoscersi soltanto all'imputato. la motivazione manca - ma lo avevo detto precedentemente - se non c'è un'autonoma motivazione dedicata ai singoli aspetti nei quali si articola il complesso della motivazione. illustri senatori, a dare delle indicazioni su alcuni aspetti più salienti: cosa in realtà rende diversa questa disciplina in maniera più pregnante

ma anche dall'articolo 311 del codice di procedura penale. Sappiamo che l'articolo 309 è regolativo della procedura dinanzi al Tribunale della libertà

all'imputato. Questa è stata una questione che ha separato l'orientamento del Senato rispetto all'orientamento della Camera dei deputati: il Senato aveva introdotto un emendamento in virtù del quale il potere di dilatare

il termine di deposito della motivazione in caso di provvedimenti particolarmente complessi). Il Senato aveva ritenuto che, anche su questo versante, endoprocessuale, *de libertate*, il collegio potesse essere facoltizzato, ossia potesse esso stesso stesso determinare, *ex officio*, una dilatazione dei tempi di deposito dei provvedimenti; la Camera dei deputati, invece, ispirata a un *favor libertatis*, aveva ritenuto che questa facoltà potesse competere solo all'imputato, il quale, se sussistono ovviamente motivi giustificativi della richiesta di dilatazione dei termini, poteva per l'appunto chiedere ed essere eventualmente autorizzato ad un sacrificio sul versante della tempestività, tempestività, che sarebbe stato eventualmente - questo nella *ratio* ovviamente non dichiarata della legge - compensato con una valutazione meno tempestiva ma più approfondita. La Camera dei deputati, quindi, ha ritenuto di tornare sul vecchio testo. Ora questa facoltà compete soltanto all'imputato; il Senato ha ritenuto di non riproporre riproporre il proprio emendamento, quindi vi è una perfetta sovrapposizione, perlomeno in questa ultima lettura, tra il testo della Camera e il testo

perentori e quelli ordinatori non differiscono in alcunché sul versante della previsione del termine, ma differiscono solo sul piano della previsione di una sanzione nel caso della loro inosservanza. Noi comprendiamo che un termine è ordinatorio esso si risolve in una sorta di consiglio, di direttiva, e non è sanzionato: io do un'indicazione ma tu sei libero di non osservarla. Certo, se vi è una sanzione, una decadenza, una preclusione, un'inammissibilità, allora apprendiamo che quel termine è perentorio. Il termine

Il termine è perentorio perché l'ordinanza cessa di avere efficacia. Noi, quindi, individuiamo la sanzione: c'è una sanzione processuale in virtù della quale l'ordinanza, perdendo efficacia, comporta la scarcerazione dell'imputato. Questo è chiaro. È pur vero che la norma consente un recupero della condizione cautelare, perché fa salvo il caso in cui esistano eccezionali esigenze cautelari che, però, devono essere specificamente motivate. Questo meccanismo decadenziale, questo termine perentorio, si recupera, non dinanzi alla Cassazione. Sarebbe, infatti, stato impossibile prevedere un meccanismo decadenziale in quel caso. All'indomani dell'entrata in vigore della normativa sul Tribunale della libertà, vi era che anche la Cassazione dovesse decidere in termini perentori, ma qualche manuale - ne ricordo qualcuno - aveva affacciato un'interpretazione coeva - potremmo dire - all'entrata in vigore, nel 1982, del Tribunale della libertà, caso era impensabile poter ipotizzare un termine perentorio. In questo caso, però, la perentorietà del termine è recuperata sul versante del giudizio di rinvio: tutte le volte in cui la Corte di cassazione, accogliendo i motivi *de libertate*, nella fase endoprocessuale del Tribunale della libertà, annulla con rinvio al Tribunale della libertà localmente collocato sul territorio, a seconda ovviamente della competenza territoriale, tale tribunale ha termini perentori per decidere nel giudizio di rinvio. Anche questa volta, con simmetria che non poteva non essere assolutamente perfetta, si stabilisce che la mancata decisione del Tribunale della libertà entro il termine perentorio determina l'inefficacia del provvedimento di custodia cautelare, sempre fatti salvi i casi di eccezionali esigenze cautelari che devono però essere specificatamente individuate. L'ultimo mio riferimento - per non disturbare troppo l'Assemblea - riguarda una norma, l'articolo 21-*ter* della legge legge penitenziaria, in virtù della quale si dilatano i permessi di visita di soggetti detenuti a vantaggio di propri congiunti. Si dilata la categoria: non sono solo i figli i beneficiari di questi permessi, ma anche i coniugi, ovvero i soggetti conviventi, purché portatori di gravi *handicap*, sia pure da stabilire sulla base delle legislazioni vigenti in materia. Mi scuso per l'eccessiva natura riassuntiva del quadro che mi sono permesso di dettare nel nel corso di questa mia relazione introduttiva. Il dibattito certamente consentirà di mettere in evidenza tutto quello che deve essere per l'appunto posto all'attenzione perché l'Assemblea abbia una perfetta conoscenza delle questioni giuridiche che questo testo legislativo pone. Comunque, io credo che gli istituti principali siano quelli sui quali mi sono permesso di richiamare particolarmente l'attenzione dell'Assemblea.

più virtuosi, che con lettera hanno già informato, attraverso l'ANCI, la Presidenza del Consiglio chiedendo con urgenza che si provveda ad emanare il decreto-legge degli enti locali. Questo decreto-legge nasce da necessità che sono state ben evidenziate in un'intesa sottoscritta proprio alla fine di febbraio nella Conferenza unificata Stato-Regioni.

lamentano, piuttosto motivatamente, che le tardive prese di posizione nel 2014 relativamente alla finanza locale

per il patto di stabilità. Ora, questo è stato evidenziato in Conferenza Stato-Regioni. Non c'è il tempo per analizzare le singole situazioni, ma credo basti affermare, alla luce di una serie di esempi che mi sono stati rappresentati da Comuni del Veneto, che che quello che purtroppo è avvenuto è che questa erronea contabilità ha, di fatto, impedito e sta impedendo loro di poter procedere con i bilanci del 2015, mettendo in campo un meccanismo che, dal punto di vista costituzionale, è in antitesi con quanto previsto sia dall'articolo 114

compensativo, che non sono stati a oggi riconosciuti ma che erano indispensabili per i 1.800 Comuni e i 30 milioni di abitanti di cui si parlava poc'anzi per evitare che questi subissero una perdita di gettato nel passaggio dal regime IMU alle aliquote TASI. L'assenza di questo importo implica di fatto

viene oggi completamente finanziato dai Comuni stessi; il che significa che ci sono Comuni che non soltanto vivono solo delle proprie risorse - e fin qui, nella situazione italiana, si può persino comprendere - ma ci sono Comuni che traggono risorse dai propri bilanci per metterle nel Fondo di di solidarietà nazionale a favore degli altri Comuni, il che è in aperto contrasto con i predetti articoli della Costituzione. Chiudo ricordando la vicenda dei Comuni montani, delle Città metropolitane e la necessità di rifinanziare il Fondo di cui trattasi. *(Applausi del

In questo modo alle lavoratrici resterebbero solo due possibilità: perdere il posto di lavoro o la ventilata possibilità di essere trasferite nelle altre aziende, che però si trovano a 350 chilometri di distanza

Negli anni della crisi non ha avuto sostanziali contraccolpi, salvo un'esperienza importante di contratti di solidarietà, per cui disporrebbe ancora di strumenti, quali la cassa integrazione ordinaria, che potrebbero garantire il superamento di un problema come come quello preannunciato riguardante una difficoltà produttiva. Purtroppo però l'azienda ha scelto un'altra strada, quella, che riteniamo gravissima, della chiusura che reputiamo immotivata, soprattutto perché immediata e lascia senza lavoro e senza futuro 230 lavoratrici in un momento in cui purtroppo la disoccupazione è ancora molto elevata anche nel territorio padovano. Abbiamo appena presentato un'interrogazione urgente al MISE. Intervengo in questa sede chiedendo alla Presidenza del Senato di farsi interprete di una risposta immediata affinché il MISE convochi immediatamente le parti per esaminare tutte le possibili alternative. Ripeto, si tratta di una produzione di alta qualità.

e hanno diritto di avere dalle istituzioni una risposta immediata e adeguata che impegni il gruppo Zegna, un gruppo prestigioso e ancora affermato nel mercato nazionale e internazionale, a recedere a recedere dalla chiusura e a trovare un'intesa sui molti strumenti che possono permettere una gestione socialmente più compatibile della situazione di difficoltà produttiva che, ripeto, può avere altre possibili

Santini, che mi ha appena preceduto, ha portato all'evidenza una problematica legata ad una questione di perdita di posti di lavoro Io invece parlerò di una problematica che tocca un po' tutto il bel Paese e che, nella fattispecie, riguarda Viterbo, qui nel Lazio. Sono stati registrati - questa ormai è storia economica degli ultimi anni - un calo dei consumi e una disoccupazione giovanile ai massimi storici, per non parlare poi di quella femminile, che in questi giorni è stata illustrata chiarezza dalla descrizione che l'ISTAT ha dato di questo fenomeno. C'è in gioco, con la perdita di questi posti di lavoro, l'equilibrio del sistema sociale di un territorio e di un intero Paese. Si è chiuso nel peggiore dei modi, secondo l'ISTAT, l'anno nero del commercio italiano: la diserzione dei negozi da parte degli italiani stessi è evidente e riguarda sia riguarda sia i prodotti alimentari che quelli non alimentari. Una sorta di*par condicio* che ha toccato la grande distribuzione e i piccoli distributori, cioè quelli che hanno delle piccole superfici. In questo contesto economico, si è svolta una manifestazione. Lo striscione che i dipendenti hanno mostrato mostrato all'universo mondo - perché le immagini sono andate sui giornali e sulle tv nazionali e locali - diceva: «Dipendenti non in svendita». dimostrazione, assolutamente pacifica, è stata organizzata per attirare l'attenzione della politica sulla possibilità sempre più concreta di chiusura del negozio della Cassia nord.

portati dalla dirigenza motivi legati al risanamento e alla ridefinizione dei punti vendita che non si sostengono economicamente. Si paventa quindi la chiusura di circa la metà dei punti vendita a livello nazionale: una sorta di di *roulette* russa, una pistola puntata alla tempia dei lavoratori, che sono circa 3.700 in tutto, di cui 1.200 sono probabilmente interessati da questo ridimensionamento o chiusura totale di alcuni punti Noi abbiamo già presentato un'interrogazione, a prima firma del senatore Arrigoni, in cui sollecitiamo il Ministero a farsi carico di questa problematica e a mettere in campo tutte le azioni per tutelare in tutti i modi i lavoratori interessati. Ieri sera abbiamo incontrato, proprio a Viterbo, una delegazione di questi lavoratori; ne mancava giusto qualcuno, ma erano ben rappresentati. abbiamo visto il grande dispiacere per la perdita di un posto di lavoro, però abbiamo visto anche la dignità che accompagna queste persone; certamente non abbiamo visto in loro la rassegnazione. Questo deve essere il sentimento che accompagna la politica, che deve mettere in campo tutto quello che è possibile fare per tutelare il posto di questi lavoratori, ma in generale anche di chi